È in corso una grande manifestazione della gente di montagna, che è venuta a Roma per protestare contro gli articoli 13 e 16 della finanziaria, affinché siano restituiti alla trattazione di una legge organica, che già è stata presentata, e siano quindi da essa stralciati. Al di là del contenuto, signor Presidente, volevo segnalare un'informazione per i miei colleghi senatori dell'opposizione. So che alle ore 13 lei gentilmente riceverà una delegazione degli organizzatori, che alle ore 13,30 si incontreranno poi con i senatori della maggioranza, e vengo alla notizia (che devo dare in questo modo e mi scuso per lo *spot* involontario): alle ore 14,30 gli organizzatori della manifestazione

Signor Presidente, ieri sera la Presidenza di turno ha deciso inopinatamente di ghigliottinare la discussione generale. generale. In un momento di confusione, senza prendere atto che molti colleghi, anche perché l'ora era tarda, si erano allontanati temporaneamente dall'Aula, con una sorta d'appello frettoloso ha di fatto privato del diritto di interloquire e di intervenire in discussione generale oltre dieci colleghi. Presidente, questo tipo di comportamento è inusuale in quest'Aula perché, in genere, quando si decideva anticipatamente di chiudere la discussione generale si convocava perlomeno

è stata presentata dal vice ministro Visco la relazione che certifica il recupero di gettito relativo all'evasione fiscale. La richiesta della sua presentazione era stata avanzata anche dal Parlamento.

e che hanno visto aprirsi un confronto serrato fra maggioranza e opposizione. L'opposizione ha affermato che si tratta di un fatto politico clamoroso perché la relazione accerterebbe che siamo di fronte al cosiddetto falso in bilancio. Eppure non si può negare che c'è un recupero, accertato dalla relazione, di 23 miliardi di euro. Si può certo negare che questo recupero derivi dalla lotta all'evasione, però bisognerebbe anche spiegare la provenienza di questi soldi. Comunque, queste maggiori risorse ci sono e sono accertate,

C'è quindi una linea comune che lega questi due provvedimenti. L'opposizione però - credo che questo sia l'elemento più interessante dal punto di vista del confronto, ed io mi concentrerò su questi aspetti

di tali problemi. C'è il finanziamento del trasporto metropolitano per le città di Roma, Napoli e Milano (800 milioni di euro); c'è un miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina (trasferimento modale da e per la Sicilia per 75 milioni); vi sono 1.075.000.000 euro per le ferrovie, per finanziare gli investimenti e la manutenzione straordinaria delle reti tradizionali (le reti che vengono utilizzate dai pendolari)

Sono interventi per incrementare le politiche sociali? Io ritengo di sì, altrimenti si spieghi quali altri interventi in questo settore dovrebbero essere adottati. una questione che è emersa ed è permanente nella discussione di queste settimane. Si dice che, anche con questo provvedimento, il Governo aumenta la spesa pubblica. Voglio ricordare che questa è una tendenza generale, che prosegue da molti anni: non è una caratteristica di questo Governo, essendolo stata anche per il Governo precedente e probabilmente in misura maggiore. La differenza è che

ha aumentato il *deficit* e il debito, mentre noi lo stiamo diminuendo (infatti c'è il dato significativo dell'aumento dell'avanzo primario). Nel 2008 cerchiamo di stabilizzare la spesa pubblica, con l'obiettivo di ridurla nei prossimi anni. Certo che è difficile, certo che questo è un obiettivo ambizioso,

Presidente, sono rimasto favorevolmente colpito da un nuovo richiamo, da una nuova aspirazione europeista dell'opposizione di centro-destra. Credo che sia un bene per tutti: per il confronto tra la maggioranza e l'opposizione e per il confronto nel Paese. Ho sentito continui richiami alla Commissione europea, alla Banca centrale europea, a EUROSTAT e ai vari istituti internazionali che si occupano di previsioni, che studiano gli andamenti dei conti pubblici nei vari Paesi, a partire dal Fondo monetario internazionale. Siamo attenti e preoccupati - lo dico in modo sereno e con grande franchezza - per alcuni

del Governo in carica; credo che questo non sia un bene e non si rende così un buon servizio al confronto nel Paese. È mio dovere, Presidente, rivolgere un richiamo all'intervento del senatore Lunardi;

sotto alcuni aspetti anche offensivo e, alla fine, astioso. Credo che ciò non vada bene perché in questo modo si dimentica il merito della questione, la soppressione degli interventi relativi allo Stretto di Messina, rispetto invece alla forma e al metodo della critica. E allora, guardate che in politica il metodo è sostanza e mi permetto, lo dico sommessamente, di rivolgere alcuni consigli al senatore Lunardi. Ritengo che la democrazia sia un esercizio complesso,

delle forze politiche che sostengono questa maggioranza e nel Governo. È quindi una scelta responsabile e approfondita: non è una scelta irresponsabile. La soppressione del progetto e la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina è stata sottoposta al giudizio dell'elettorato, che ha premiato questa coalizione, di poco, ma l'ha premiata: è inutile non ricordare questo aspetto. Forse, il senatore Lunardi se ne è dimenticato, però è un male innamorarsi dei propri progetti perché, alla fine, chi decide non è solo la politica, la politica, ma l'elettorato in modo democratico. Se non si capisce questo, si parla al vento mentre la politica si sta occupando di altro. C'è un altro. C'è un ultimo aspetto che non posso dimenticare. Il senatore Lunardi ha rivolto critiche abbastanza pesanti, persino offensive, nei confronti dei ministri Bianchi

Critiche offensive nei confronti dei ministri Bianchi e Pecoraro Scanio; due Ministri, ha detto il senatore Lunardi, che hanno fatto prevalere la forza dell'ignoranza.

Ritengo di essere una persona tollerante e cerco di comprendere le ragioni dei miei avversari. Le ragioni di chi ha sostenuto quel progetto, al di là degli insulti, sono molto deboli.

intervenendo ripetutamente per consentire ai Ministri di raggiungere l'Aula del Senato), abbiamo appreso, anche con una certa soddisfazione, che era stato approvato dal Consiglio dei ministri il pacchetto sicurezza. Il ministro Pecoraro Scanio, uscendo dal Consiglio dei ministri, non solo aveva annunciato che era stato approvato il pacchetto, ma era anche entrato nel merito, facendo degli apprezzamenti su alcuni articoli che erano stati approvati; addirittura, era molto contento perché era stato approvato un articolo che inaspriva le pene per coloro che provocano incendi. Ieri sera mi sono fatto immediatamente partecipe: ho telefonato a Palazzo Chigi per cercare di avere il testo del pacchetto sicurezza che era stato approvato ed ho ricevuto una risposta molto imbarazzante.

Mi sembra giusto ed opportuno che l'Assemblea del Senato sappia cosa è accaduto in quel Consiglio dei ministri molto travagliato.

La dignità del Parlamento e del Senato (mi rivolgo anche a lei, senatore Matteoli, perché ha sollevato la questione), a mio avviso, si difende anzitutto non parlando di acquisto di senatori, ma svolgendo una puntuale attività parlamentare, così come hanno fatto, insieme al Governo, i senatori della Commissione bilancio, che ha esaminato e sviscerato ogni norma di questo decreto, migliorandone alcune ed aggiungendone altre. Ringrazio perciò tutti i componenti della Commissione, che hanno lavorato molto e bene. Do atto ai senatori dell'opposizione del loro contribuito, che in molti casi è stato considerato dal Governo, con l'accoglimento di molti emendamenti dei Gruppi di opposizione. Naturalmente, il mio ringraziamento va al relatore e al Presidente della Commissione: il loro lavoro è stato prezioso e proficuo. In un momento di imbarbarimento della politica e di accentuata antipolitica, considero un dato positivo il fatto che in Commissione bilancio vi sia stata una corretta dialettica politica; anche in quest'Aula, al di là di un singolo intervento che ritengo fuori dalle righe, il dibattito è stato interessante e ringrazio quanti hanno ritenuto di intervenire su un provvedimento complesso, ma che è parte corposa dell'intera manovra finanziaria del Governo. Indubbiamente, la discussione sul decreto-legge n. 159 non poteva non allargarsi all'intera manovra finanziaria presentata dal Governo; questa, oggettivamente, va valutata anche alla luce dei mutamenti economici a livello mondiale. L'economia italiana - come ha ricordato il senatore Bonadonna - subisce i riverberi del contesto internazionale. La crisi finanziaria determinata dai mutui *subprime* negli USA ridisegna la mappa economica mondiale, rallenta la fase espansiva negli Stati Uniti e i Paesi cosiddetti emergenti acquistano un peso sempre più rilevante nella crescita globale. Il Fondo monetario internazionale stima che il peso della Cina, dell'India e della Russia è ormai del 50 per cento. Ovviamente, ciò non può che incidere sull'economia dell'eurozona e dell'Italia, sull'*export* del nostro Paese. Negli Stati Uniti e in Inghilterra vi sono state preoccupanti manifestazioni dei risparmiatori, ma anche in Italia i prodotti derivati e i mutui variabili hanno creato non pochi problemi, soprattutto alle piccole e medie imprese e ad alcune Regioni ed enti locali. In merito, la senatrice Bonfrisco ha presentato un emendamento che, se riformulato, sarà accolto dal Governo, che comunque segue la vicenda con grande attenzione. L'anno scorso la manovra finanziaria che, ricordo, fu di ben 35 miliardi - fu improntata in misura preponderante al risanamento dei conti pubblici; gli effetti si sono avuti e i dati sono eloquenti, senatore Ciccanti. Certo, occorre proseguire su questa strada; è nostro dovere farlo, perché il debito pubblico è davvero enorme. Però, i dati, al di là delle polemiche, sono davvero chiari. Ricordo a me stesso che l'avanzo primario è passato dallo 0,1 del 2006 al 2,5 del 2007, il rapporto *deficit*-PIL si è ridotto dal 4,4 del 2006 al 2,4 del 2007. Come già riportato nel Documento di programmazione economico‑finanziaria e nella Nota di aggiornamento, le misure *una tantum* nel 2006 hanno inciso per l'1,2 sul PIL; pertanto, al netto il disavanzo è stato pari al 3,3 Facendo lo stesso calcolo per il 2007, si stima un disavanzo pari al 2,5, incidendo per lo 0,1-0,2 le misure a carattere straordinario. In pratica, l'indebitamento netto tra il 2006 e il 2007 si è ridotto e le entrate sono aumentate. Si può discutere, senatore Baldassarri, su quanto abbia inciso la lotta all'evasione, ma è innegabile - come risulta dalla relazione presentata, anche se in ritardo che tra il 2006 ed il 2007 sono stati recuperati al fisco circa 23 miliardi di maggiori entrate: dati certi, non falsati.

A luglio si fece una operazione di 0,4 punti di PIL, si redistribuì il primo extragettito, determinato dal recupero di base imponibile, dalla lotta all'evasione e, per un terzo, dall'andamento dell'economia. La manovra finanziaria attuale è profondamente innovata nella sua struttura. Mi rivolgo alla senatrice Valpiana, che ha posto questo problema ieri sera. La modifica, ancora non sufficiente, è merito anche del contributo delle Commissioni parlamentari del Senato e della Camera.

Il nesso è determinato dal fatto che esso dà attuazione ad importanti interventi previsti nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. Trattasi di oneri derivanti dal contratto del pubblico impiego, dagli accordi per la cooperazione internazionale e dagli interventi per le ferrovie e l'ANAS.

tutte le risorse disponibili derivanti dalle nuove entrate ad un'ulteriore riduzione del debito pubblico. Le condizioni economico-sociali e territoriali del nostro Paese non consentono una scelta drastica, *tout* *court*, di tale portata. Il Governo non sarebbe né responsabile, né coerente con il programma presentato se, dopo aver ridotto in misura notevole il rapporto *deficit**-*PIL ed inciso, anche se di poco, sull'ammontare complessivo dell'indebitamento, non intervenisse a sostegno delle fasce più deboli della nostra società e dello sviluppo complessivo del Paese. Le scelte riguardano anche il taglio della spesa. Il Governo ha scelto, perciò, un percorso rigoroso, ma graduale. di legge finanziaria si prevede una riduzione della spesa corrente con provvedimenti incisivi, che non riguardano soltanto il numero delle comunità montane e la riorganizzazione degli uffici e quant'altro.

8.321 milioni di euro: in parte, allo sviluppo e alle infrastrutture, alla ricerca e all'innovazione; in parte, ripeto, alle fasce più deboli. Non credo che destinare risorse all'ANAS, alle Ferrovie, alle metropolitane di Milano, Roma o Napoli, all'edilizia abitativa pubblica, alla costruzione di terminali di rigassificazione possa assumere il significato di uno spreco, di un gettare ulteriori risorse in un pozzo senza fondo. Significa, invece, creare ricchezza collettiva e condizioni per accelerare la crescita economica del Paese, aumentare la vivibilità nei vari territori e, soprattutto al Sud, l'*appeal* per gli investitori. Gli stessi interventi destinati agli incapienti e al rinnovo dei contratti, oltre a dare un minimo di sollievo alle famiglie dei lavoratori, non potranno che fare bene all'economia, incidendo soprattutto sui consumi. Perciò, senatore Curto, nessun passo indietro sulla strada del risanamento, dello sviluppo e dell'equità, intrapreso con il primo provvedimento Bersani, con la finanziaria 2007 e proseguito, con coerenza e tenacia, prima con il decreto-legge n. 81 del luglio scorso ed ora con questo decreto-legge. Il senatore Ferrara, con la sua solita puntualità argomentativa, ha sostenuto il non rispetto della legge di contabilità e degli accordi con l'Europa. Come evidenziato nel *dossier* del Servizio del bilancio del Senato, gli effetti complessivi del decreto-legge, senatore Ferrara, non stravolgono gli obiettivi concordati in sede europea,

Il Governo, perciò, rivendica la positività delle scelte di fondo di questo decreto. Destinare una parte significativa delle risorse agli incapienti è un dovere, politico e morale. Certo trattasi di somme individuali esigue, ma non di mance, senatore Curto, perché quando si concede anche un solo euro a chi è indigente lo si deve fare con rispetto. E noi verso queste fasce deboli abbiamo il dovere, tutti, di essere rispettosi. Certo, è poco. Vorremmo e dovremo fare di più, ma non c'è bisogno di richiamare proverbi cinesi, come ha fatto il senatore Ciccanti, al quale ricordo che dalle mie parti, in Basilicata, nel Mezzogiorno, c'è un altro proverbio, che dice che chi è sazio non crede a chi è digiuno. Perciò anche poco è meglio di niente. Purtroppo in passato gli incapienti non hanno avuto niente. L'intervento del senatore Lunardi è stato poi particolarmente tagliente e bene ha fatto il relatore a ricordarlo. È stato tagliente nell'attribuire al Governo comportamenti terzomondisti e una cultura intrisa di un integralismo sinistro che non ci appartiene. Si può criticare la scelta di sopprimere la società Stretto di Messina, ma non ci si può accusare di non pensare allo sviluppo e alle infrastrutture del Mezzogiorno, in Sicilia e in Calabria. Anche in questo decreto vi sono risorse destinate a tale scopo. E comunque, per quanto riguarda questa scelta, essa è compiuta in sede parlamentare, perché il Governo si è rimesso, nel caso specifico, alla volontà del Parlamento. si può stare tranquilli che il decreto non sconvolgerà i conti pubblici ed è coerente con la complessiva politica economica del Governo. È un decreto che, insieme alla finanziaria, non toglie alle famiglie, ma dà; non aumenta le tasse, ma restituisce qualcosa, soprattutto ai più deboli. Ha ragione la senatrice Pellegatta quando afferma che occorre rafforzare il senso dello Stato e dell'etica, puntando sulla cultura e sulla conoscenza per avere più senso della comunità, della collettività. Questo Governo, fin dal suo insediamento, si è mosso e ha agito nella consapevolezza di elevare la quantità e la qualità dello sviluppo, cui anche questo decreto finalizza alcune risorse, non soltanto per dare ai nostri concittadini migliori condizioni di vita e di lavoro, ma per tutelarne e garantirne i diritti e ridare al nostro Paese quello slancio morale ed ideale che fa grande una Nazione del mondo.

In sede di esame del provvedimento in titolo, sono emerse una serie di contraddizioni relative anche alle disposizioni dell'articolo 12. dove si parla di sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione, si aumentano di 150 milioni di euro i fondi disponibili per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione disposto dalla legge finanziaria per bloccando l'operatività della clausola di salvaguardia, con l'effetto di rallentare il processo di riduzione del personale. I rischi connessi alla mancata applicazione della clausola di salvaguardia, recata dall'articolo 1, comma 621, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, sono sono confermati negli stessi documenti di bilancio per il 2008, che pongono l'attenzione sul peggioramento dell'indebitamento netto di circa il 50 per cento a fronte delle minori economie conseguite nell'anno medesimo. Al riguardo, si precisa che il comma 621, lettera *b**)*, della legge finanziaria 2007 non prevedeva né una sua applicazione parziale né, conseguentemente, risparmi inferiori a 448,2 milioni di euro per l'anno in corso. L'assegnazione integrativa per il 2007 non è giustificata dal carattere di eccezionalità e, in specie, sarebbe altresì utile conoscere i criteri che si intende applicare per la predetta integrazione, a valere sugli anni successivi all'anno in corso. Il Governo, peraltro, sostiene l'adempimento dell'obbligo scolastico ridefinito al comma 622 della legge del 23 dicembre 2006, n. 296, contravvenendo ancora una volta alle regole che non consentono di inserire nell'ambito di una manovra finanziaria norme di delega o di carattere ordinamentale, ovvero organizzatorio, nonché violando le competenze di carattere normativo attribuite alle Regioni dalle disposizioni costituzionali, nel richiamato articolo 117, terzo comma, della Costituzione, senza tener conto del parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni, anche in considerazione di eventuali contrazioni delle attuali competenze regionali in tema di istruzione e di formazione professionale. L'estensione dell'obbligo scolastico al di là dell'istruzione inferiore è incostituzionale, salvo che il legislatore non qualifichi anche il biennio delle attuali scuole superiori come facente parte dell'istruzione inferiore. Tutto ciò premesso, avanzo la proposta di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1819, così come previsto dall'articolo 96 del Regolamento del Senato.

In particolare, ritiriamo gli emendamenti: 7.15, 8.17, 8.0.2, 10.15, 14.0.6, 19.0.1, 21.6, 26.0.800/2,

Signor Presidente, intervengo per motivare politicamente, più che tecnicamente, il nostro voto contrario alla richiesta di non passaggio agli articoli proposta dal Gruppo della Lega Nord Padania. Il non passaggio agli articoli, in effetti, sembra più che altro reiterare un insistito tentativo dell'opposizione di mettere in difficoltà la maggioranza su questioni procedurali. In ogni seduta dei nostri lavori, i colleghi della minoranza si esercitano con tentativi - a volte anche sofisticati e raffinati, altre volte un po' più grossolani - per costellare di ostacoli più o meno artificiali il già arduo cammino della maggioranza. È naturalmente fuori discussione la legittimità di questa battaglia tecnico-formale, ma, se mi è concesso di parlare con franchezza, in alcuni casi l'insistenza con la quale viene proposta e riproposta appare più il frutto di un'ostinata volontà a riproporre uno schema fisso di lotta parlamentare piuttosto che di rispondere ad ad un progetto politico di più ampio respiro. Nel caso in discussione, soprattutto, questa richiesta sembra un sovrappiù rispetto alla discussione che ci attende sulle centinaia di emendamenti presentati, nonostante gli ultimi ritiri testè annunciati. Vorrei richiamare tutti noi al grande senso di responsabilità dimostrato in primo luogo dalle forze dell'opposizione in Commissione bilancio, laddove è stato possibile, grazie a quello stesso senso di responsabilità, esaminare nel dettaglio tutto l'articolato, tutti gli emendamenti, raccogliere, in diversi casi, gli stimoli positivi e le proposte della opposizione. Senso di responsabilità che permette oggi all'Aula di discutere ancora, nel merito, le proposte nuovamente presentate all'attenzione di tutti i colleghi e le colleghe.

si parte al rallentatore: c'è un tentativo di mettere in difficoltà la maggioranza. Mi auguro che nel prosieguo dei nostri lavori prevalgano quello spirito di responsabilità quella volontà di corrispondere alle attese del Paese, ragionando in maniera responsabile su un disegno di legge che, in qualche modo, risponde a criteri di urgenza e a bisogni impellenti dell'Italia. Mi auguro quindi che, superato anche questo voto, si possa entrare nel merito delle singole proposte ed arrivare speditamente all'approvazione del disegno di legge in

dopo avere ascoltato con un po' di meraviglia la relazione del collega Ripamonti,

In poco più di un anno, sottosegretario Lettieri, come le ricordavo ieri sera, il gettito tributario è aumentato di 45 miliardi. Se si considera l'aumento degli oneri sociali di 15,7 miliardi - che saliranno di altri 10 miliardi nel 2008 il complesso delle entrate, come ricchezza sottratta al Paese, ammonta a 65 miliardi, di cui la metà è stata da voi destinata a maggiori spese. È su questi dati che dovete riflettere: si tratta di ben 4,3 punti di PIL. Se le maggiori entrate registrate fossero state destinate alla riduzione del disavanzo, questo oggi si attesterebbe all'1,5 per La Nota di aggiornamento al DPEF presentata dal Governo, invece, ha rivisto gli obiettivi di indebitamento netto per il 2007 al 2,5 sicuramente inferiore al 2,8 deciso a livello ECOFIN, su cui vi state nascondendo, ma con un differenziale superiore certamente allo 0,5 per cento, previsto in sede ECOFIN, per il rientro nel pareggio di bilancio nel triennio 2008-2010. Si tratta di stabilire se si rende un servizio alla comunità nazionale rimandando alle future generazioni un debito tra i più alti d'Europa; oppure, riducendo oggi la spesa pubblica corrente, intendendo escludere, ovviamente, la spesa sociale, che va ristrutturata in modo da non dare tutto a tutti, ma solo a chi ha veramente bisogno. In questo senso intendiamo privilegiare la spesa in conto capitale, quella degli investimenti sulle infrastrutture, perché riguarderà le future generazioni. Questo è il dovere morale e politico di una classe dirigente. Sosteniamo perciò tutti gli emendamenti che vanno in tale direzione nel decreto-legge dell'UDC, comunque, intendiamo sfidare la maggioranza e il Governo annunciando che ritireremo tutti i nostri emendamenti se il Governo e la maggioranza rinunciano alla spesa del tesoretto, ripartito nel decreto-legge n. ferma restando ovviamente la spesa sociale per gli incapienti e le infrastrutture strategiche di rilievo nazionale. Vedremo se sarete bravi ad accettare la nostra sfida. Signor Presidente, prendo la parola per indicare all'Aula l'opportunità di votare contro la proposta di non passaggio agli articoli.

Quand'è che si procede al non passaggio agli articoli? Quando si vuole impedire che la trattazione dell'argomento prosegua e questo può avere motivazioni tecniche o politiche; può darsi che la materia non sia stata correttamente affrontata, che non sia stata adeguatamente approfondita. In questo caso, invece, credo sia evidente la motivazione politica che sta dietro la proposta dei colleghi dell'opposizione, che si trovano nella difficoltà che non può essere dichiarata ma tuttavia, a mio modo di vedere, è evidente - di essere di fronte ad un'iniziativa del Governo e della maggioranza che, diversamente da quanto ieri è stato detto, non mette affatto le mani nelle tasche degli italiani ma al contrario mette qualcosa nelle tasche degli italiani. Ritengo che sia stata evidente questa natura nel corso della discussione in Commissione e anche adesso nei primi approcci di Aula. Abbiamo un'iniziativa che si affianca al disegno di legge finanziaria e che comincia a dare nell'insieme il segnale di un'azione di Governo che esce dalla fase emergenziale che ha connotato il primo avvio dell'esperienza in questa legislatura del centro-sinistra e comincia a dare risposte più vicine ad un assetto definitivo. È un'iniziativa che politicamente assume il segno di un avvio di normalità, di un'azione di Governo che non risponde alla necessità immediata e pressante di rimettere in sesto i conti pubblici. Tale iniziativa prende atto che il primo contrasto,

dunque, in questo decreto, e poi con la finanziaria, c'è una nuova attenzione alla distribuzione di risorse che si rendono disponibili, con l'inizio di un'azione di Governo complessivamente attenta

in qualche modo ridurre il dubbio della costituzionalità, che alcune delle norme contenute nel decreto potevano e possono fare nascere.

alla richiesta di non passaggio agli articoli. Comprendo perfettamente che la manovra che si sta mettendo in campo, tra questo decreto e la finanziaria, possa essere per i colleghi dell'opposizione un elemento di preoccupazione politica. Segna, infatti, un cambio d'indirizzo, che andrà perfezionato e approfondito, ma che, dal loro punto di vista, rappresenta un rischio per l'esito politico di quanto il Governo e la maggioranza stanno mettendo in campo. esattamente questo stesso motivo - rovesciato - che induce la maggioranza a sostenere, invece, la necessità che l'*iter* di formazione di quest'atto prosegua e che quindi esso sia discusso in quest'Aula,

un pezzo molto significativo della complessiva azione del Governo nell'attuale fase. Contribuisce - come ho detto - a determinare un primo, corposo e importante segnale al Paese del cambiamento, cambiamento, di una nuova attenzione e di una nuova fase dell'azione di Governo, che è consentita, resa possibile e

un'operazione politica i cui contenuti sono in totale contraddizione con gli obiettivi annunciati. Quindi, delle due l'una: o Governo e maggioranza stanno compiendo una mistificazione nei confronti del Paese oppure la maggioranza non ha ben compreso cosa il Governo propone.

I numeri ai quali lei fa riferimento sono quelli sbagliati comunicati dal Governo Amato alla Commissione europea e all'EUROSTAT e corretti due anni dopo dallo stesso EUROSTAT. I numeri veri sono quelli

ci mancherebbe, visto che le mani in tasca agli italiani le avete messe per oltre 45 miliardi di euro (con il decreto Visco-Bersani per 7 miliardi,

nascosto, come ben noto e dimostrato dalla relazione comunicata in grave ritardo dal Governo ieri al Parlamento, 23 miliardi di euro che a tutt'oggi non sono neanche stati contabilizzati, visto che nella Nota di variazione al DPEF ne avete inseriti solo 19. Quindi, gioco delle tre carte e trucchi contabili, con il risultato di avere una maggiore pressione fiscale (dal 40,6 al 43,1 per cento), una maggiore spesa pubblica corrente accentrata nei Ministeri, Ministeri, a scelta discrezionale dei Ministri, e un maggiore *deficit* pubblico, che la Banca d'Italia ha certificato essere quest'anno attorno all'1,5

il*deficit* pubblico, che nei dati tendenziali, senza le vostre manovre, sarebbe quest'anno dell'1,2

o maggioranza e Governo sono consapevoli di quanto fanno e quindi in contrasto con i loro obiettivi, perché si frena lo sviluppo, si aumenta il *deficit* pubblico e non si fa equità sociale (con 41 miseri centesimi al giorno agli incapienti come *una tantum,* 81 miseri centesimi al giorno alle pensioni minime

e quindi sono consapevoli di mistificare il messaggio all'opinione pubblica e cioè di dire che si assumono provvedimenti per lo sviluppo, il risanamento e l'equità sapendo sta frenando lo sviluppo e aumentando il*deficit* senza fare equità fiscale e sociale, oppure occorre che la maggioranza rifletta, legga i documenti del Governo e si renda consapevole che quanto sta per approvare è un decreto che disperde le risorse a pioggia, non aiuta i deboli, frena la crescita e aumenta il *deficit* pubblico. Lo avete già fatto con il decreto

che determinerete quest'anno e l'anno prossimo, dal quale andrà sottratto parzialmente quel tesoretto che state nascondendo e preparando per il 2008.

cioè un nuovo gettito oggi costruibile e calcolabile, non contabilizzato, così da poter pronunciare ancora una volta la più clamorosa delle menzogne, e cioè che nascondendo i numeri e facendoli emergere qualche mese dopo si fa la lotta all'evasione. Francamente, c'è molta tristezza in queste mie parole ma ci dovrebbe essere un pizzico di vergogna da parte della maggioranza e del Governo. *(Applausi dai Gruppi AN e

reca una reintegrazione del fondo destinato all'istruzione per coprire il conseguimento parziale dell'obiettivo di riduzione del personale ATA. all'Aula che la legge finanziaria del 2006 prevedeva in un anno solo un obiettivo, troppo ambizioso, di riduzione di questo personale di 43.000 unità, che esso è stato conseguito solo in parte per 14.000 unità, ma che a tale obiettivo non si rinuncia nel triennio poiché l'aggiornamento contenuto nel disegno di legge finanziaria

che porta ad un effettivo risparmio in questo comparto di spesa. Credo che tutto possiamo dire ma non che il Ministero dell'istruzione sia stato sia stato poco attento alle esigenze di razionalizzazione e di riduzione della spesa. Il conseguimento di un obiettivo di tal genere in così poco tempo

e cioè a bloccare l'operatività di questo decreto sulla scorta delle argomentazioni testé svolte dal senatore Baldassarri e prima ancora dal senatore Ciccanti che meritano alcune argomentazioni di contrasto.

manovre in corso d'anno che hanno provveduto ad una utilizzazione virtuosa dell'extragettito che si è determinato, sia

più nel dettaglio, nel famoso comma 4 della legge finanziaria per il 2007, ma per finalità di altro tipo, criteri di interventi a pioggia, dissipazione di denaro. Basta esaminare attentamente il contenuto dei due provvedimenti - in particolare quello di cui stiamo discutendo - per trarre argomenti solidi circa la totale infondatezza e la pretestuosità degli argomenti che sono stati al riguardo spesi. A me preme sottolineare un ulteriore dato, e cioè che si assume i saldi peggiorano. Non comprendo come si possa sostenere una tesi del genere se si considera che il risultato del combinato della manovra finanziaria dello scorso anno, dei due decreti e della manovra di bilancio di cui discuteremo nei prossimi giorni è quello di un netto miglioramento dei saldi rispetto agli obiettivi concordati in sede europea. Si sostiene che potevamo fare di più. E certo che potevamo fare di più. Si sostiene che potevamo accelerare sul piano del risanamento. E certo che potevamo accelerare sul piano del risanamento. Ma si può sostenere questa tesi e al contempo dire che si fa poco per le infrastrutture, per l'equità e per la riduzione della pressione fiscale? Non si possono sostenere queste tesi tutte insieme. Mi sembra un'ovvietà.

il risanamento, lo sviluppo e la crescita -, oppure non si regge la politica economica e finanziaria del Governo. Dal momento che noi crediamo che questa politica sia quella di cui il nostro Paese ha bisogno, riteniamo che al verificarsi del miglioramento delle entrate (e comunque, in generale, delle condizioni della finanza pubblica) debba conseguire

determinano, in combinazione con il rilevamento dell'extragettito, un miglioramento dello 0,4 per cento rispetto al dato di indebitamente netto programmato:

La verità è che queste misure non corrispondono compiutamente agli obiettivi che noi vorremmo porci sul tema dello sviluppo e dell'equità sociale.

e previsti, ma non sono neanche lontanamente comparabili a quelli che furono conseguiti nel quinquennio di Governo del centro-destra. Ricordo all'Aula che il rapporto *deficit*-PIL nel 2002

Nel 2004, dal 2,2 programmato si arrivò al 3,5; nel 2005 dal 2,7 al 4,2. Ma vogliamo parlare, come avete fatto voi, dell'andamento dell'avanzo primario, questa speciale forma di accumulazione che con il nostro Governo è tornata a crescere a ritmo sostenuto (ricordo che la Nota di aggiornamento al DPEF prevede che si assesti al 2,7 per cento nel corrente anno e al 2,9 per cento nel 2008)? Ebbene, nel vostro quinquennio l'avanzo primario è sceso da un solido 5,3 del 2001 allo 0,1 per cento nel 2006; avete divorato il risparmio che era stato accumulato con le politiche degli anni trascorsi. tuttavia, un altro argomento che viene speso a sostegno del blocco, dell'asserita erroneità ed inefficacia di queste manovre

e che, quindi, il Governo non avrebbe fatto fino in fondo chiarezza sui conti, sulla natura e sul carattere permanente ovvero strutturale delle entrate. Su questo punto, abbiamo da ieri una novità importante: una novità importante: la relazione rimessa dal Governo, dal vice ministro Visco, sui risultati della lotta all'evasione, sull'esatta individuazione sull'esatta individuazione della natura dell'extragettito e sulla qualificazione del suo carattere permanente e strutturale; ma su questi argomenti torneremo nel prosieguo della discussione

l'emendamento 1.2 serve a riportare l'azione del Governo in materia di politica fiscale al contenuto della finanziaria del 2007. Secondo la finanziaria, le eventuali maggiori entrate dovrebbero essere utilizzate per la riduzione della pressione fiscale e tale dovrebbe essere lo scopo di questo inutile decreto. Invece questo decreto-legge, che credo sia dettato da null'altro che dalla paura di perdere le prossime elezioni, dispone spese a pioggia senza rendersi conto che in realtà si dovrebbe fare un'azione di contenimento della spesa pubblica e migliorare i saldi ovvero, come vorrebbe la finanziaria, restituire le imposte pagate in più dai contribuenti. Questo decreto‑legge non lo fa, anzi dispone una serie di spese, per cui francamente sarebbe meglio non passare neanche all'approvazione del decreto o comunque ritornare alla base di ciò che era stato fatto. Ieri è stato diffuso un documento, francamente imbarazzante, del Ministro o del Vice ministro dell'economia e delle finanze, sui risultati della lotta all'evasione. È un documento che nella prima pagina sembra un riassunto di quello che avrebbe potuto fare un Ministro della cultura popolare della stampa e propaganda di regime, perché si dicono cose che non hanno alcun senso, tant'è vero che nella parte poi dove si spiega la politica fiscale si smentiscono le premesse politiche. Si assumerebbe che in questo Paese esiste una enorme evasione e che i cittadini, da quando esiste il radioso Governo di centro-sinistra, sono lieti di pagare le tasse, perché forse hanno paura di non adottare questo comportamento; poi si spiega che il gettito è aumentato semplicemente perché le misure non antielusive, ma di spremitura (soprattutto dell'impresa), hanno funzionato. Grazie, era facile. Detto questo, visto che la pressione fiscale è salita di due punti nell'ultimo anno, bisognerebbe invece tornare ad una pressione fiscale più ragionevole, ad un rapporto più civile

con riferimento ai singoli contribuenti, sia con riferimento alla necessità di consentire di disporre di maggiori risorse per poter procedere ad uno sviluppo un po' meno stentato stentato del Paese. Per questi motivi, l'emendamento mira a riportare la questione, a rimettere sui piedi ciò che fino adesso era capovolto sulla testa e a far sì che venga veramente applicato il comma 4 dell'articolo 1 della finanziaria, restituendo ai contribuenti, per via di una minore pressione fiscale, il maltolto sottratto da questo Governo che, anziché prevedere misure di contenimento della spesa, anziché ascoltare quello che dicono importanti organismi internazionali a tutti i livelli (dal Fondo monetario all'Unione Europea), ma anche raccomandano organismi interni (come ad esempio la Banca d'Italia), dunque anziché migliorare e contenere la spesa pubblica diminuendo la pressione fiscale si dà alla spesa facile. Caro siamo tornati, alla politica di Agostino Magliani, a quella della spesa facile, ma questo non fa bene al Paese e neanche a chi la sta disponendo attualmente, perché giustamente i cittadini non gradiscono e si rivolteranno contro una politica di questo tipo, che spreca le loro risorse per

interverrò molto brevemente. Di fronte a queste entrate fiscali che vengono, per così dire, sperperate in mille rivoli, noi abbiamo posto il seguente problema. Ci sono Ci sono 4,8 milioni di contribuenti che devono ricevere dall'amministrazione finanziaria 24,4 milioni di euro, 10,9 dei quali a rischio prescrizione,

che hanno sollecitato tali rimborsi. Crediamo che questa proposta sia un atto di giustizia per evitare che queste norme di risorse fiscali vengano prescritte.

un tema straordinariamente attuale, come quello relativo ad una diversa tassazione delle componenti variabili del salario - come sono gli straordinari, i premi, gli incentivi, le liberalità

dell'aliquota applicata alla persona nel precedente biennio). In questo modo si incoraggia il rapporto tra il salario, la maggiore produttività del lavoro e la maggiore competitività dell'impresa. Ragionevolmente l'onerosità dell'emendamento è largamente compensata dall'emersione di molti di molti redditi che oggi sono in parte inevitabilmente sottratti alla tassazione perché le parti frequentemente possono colludere nel pagamento in nero di queste prestazioni, stante l'altissimo livello livello della pressione fiscale e il definirsi quindi di aliquote marginali proprio in relazione a redditi più virtuosi, come sono appunto quelli che si collegano ad esigenze di flessibilità organizzativa o di maggiore produttività del lavoro nell'impresa.

anche nel dibattito tra le organizzazioni sindacali, che è quello di intervenire sulla tassazione degli

Signor Presidente, ha fatto bene a parlare di "Governi" al plurale: è un *lapsus* nel senso che magari, nei prossimi mesi, avremo modo di trovarne un altro. Questo Governo sicuramente ha la memoria corta. Giustamente il collega Legnini ha cercato di tamponare la

entrate, a carattere permanente, dovessero essere destinate prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e, in secondo luogo, alla riduzione della pressione fiscale

Avevate l'obbligo, lo avete dichiarato, di restituire quei soldi ai cittadini e, prima di tutto, a chi paga. Noi ricordiamo

la tanto decantata evasione del Nord se sull'IRAP, in termini medi, abbiamo una evasione massima, dichiarata poi nella tabella,

**Il Senato non approva.**

del DPEF. Non era un ordine del giorno, ma un emendamento con cui si impegnava il Governo a prevedere un ridimensionamento della compagine governativa con particolare riferimento riferimento ai Sottosegretari. Correttamente, il relatore ha parlato dell'autonoma potestà del Presidente del Consiglio in relazione al numero dei Ministri, pochi giorni fa abbiamo letto una dichiarazione del Presidente del Consiglio in cui egli affermava che il numero dei Ministri dipendeva invece da una scelta dell'onorevole Fassino e dell'onorevole Rutelli e quindi questa potestà non è stata In questa sede, numerosi esponenti anche di rilievo avevano espresso il loro accordo rispetto alla proposta, ma avevano giudicato non competente la sede in cui si andava a ridiscutere, cioè quella dell'esame della

in sede di Commissione quegli emendamenti sono stati dichiarati inammissibili; la stessa inammissibilità verrà dichiarata anche rispetto agli emendamenti riproposti in Aula, per disomogeneità della materia. Cosa ci sia di omogeneo in questo decreto mi sembra difficile trovarlo, comunque posso accogliere questa valutazione e giudicare condivisibile l'inammissibilità. però quest'Aula ha veramente la volontà di dare un indirizzo al Governo rispetto al sovradimensionamento del suo organico (ricordiamo che questo è il *record* storico della storia della Repubblica), se si dovrà discutere in sede di legge finanziaria, dovremo esprimerci con un ordine del giorno dando appunto un indirizzo. Può darsi che quest'Aula sia contraria al fatto che quel sovradimensionamento sia eccessivo e che debba essere confermato, ma con questi temi aperti sui costi della politica è bene che ciascuno si assuma la responsabilità di se giudica conforme al momento storico la presenza di un Governo di 103 elementi. Purtroppo, sappiamo benissimo che questa impossibilità a procedere non è dettata da una volontà, ma dall'impossibilità di farlo, perché molti di essi sono stati dimissionati e non certo spontaneamente anche da queste Assemblee e hanno perso la carica di deputato o senatore e oggi si verificherebbe il fatto incredibile di dover dimissionare qualcuno che era stato prima costretto a dimettersi nonostante la volontà espressa dagli elettori. Chiedo quindi un voto a sostegno di questo ordine del giorno, senza nascondersi più dietro ai giochini: se si vuole ridurre il numero dei rappresentanti del Governo, si vota a

Una tecnica di diniego dell'ammissibilità degli emendamenti che fa sì che sempre siano rinviati ad un'altra sede credo che debba finire, quindi penso sia giusto condividere quest'ordine del giorno e affrontare la materia direttamente, se non qui, certamente nella discussione

Signor Presidente, il mio voto su quest'ordine del giorno sarà conforme all'orientamento del relatore. Volevo approfittare però dell'occasione fornita dalla presentazione di quest'ordine del giorno per informare l'Aula - poiché si tratta di un tema di grande rilievo politico - dell'orientamento che esplicitamente ho già annunciato in Commissione bilancio a proposito degli emendamenti che riguardano questa materia.

di ripristinare in vita - lo dico adesso in maniera sbrigativa - la legge Bassanini sulla struttura del Governo. Quegli emendamenti al decreto

l'Aula sarà impegnata nella votazione degli emendamenti alla finanziaria a distanza di dieci giorni, penso che sia la soluzione migliore rinviare a quella sede, dove potremo pronunciarci su emendamenti

spero che la proposta del relatore venga accolta e che, in questa sede, si voti contro quest'ordine del giorno, per affrontare il tema, ripeto, in modo risoluto sugli emendamenti che sono stati presentati in proposito.

proprio perché impegna da subito Parlamento e Governo nei sensi e sulle linee indicate dal presidente Morando. Il collega Calderoli ha già ricordato

verrà discusso in sede di legge finanziaria: è un ordine del giorno e rafforzerebbe quell'opinione. Capisco l'imbarazzo che può avere la maggioranza nel votare un ordine del giorno con questo contenuto poiché, come abbiamo visto tutti, dal 14 ottobre c'è un Presidente del Consiglio che rivendica *pro tempore* la potestà di decidere il numero dei Ministri e c'è un altro Presidente del Consiglio, *in pectore*, che invece invita il Presidente del Consiglio *pro tempore* a tagliare a metà il numero dei Ministri.

la menzogna inizia ad essere ripetuta e questo pomeriggio avrò modo di parlare delle menzogne soprattutto quando vengono da una certa Commissione. non sono un disposto normativo; sono un atto di indirizzo rispetto al Governo e alle posizioni che dovrà assumere in sede di Commissione e poi in Aula. Il fatto di voler votare contro la riduzione dei rappresentanti del Governo sta a significare che questa Assemblea, questi senatori non vogliono che vengano ridotti i numeri. Così come nel successivo,

e le richieste che ci vengono dall'Europa. Quindi o c'è la volontà di impostare un contenimento della spesa pubblica, e lo si deve dimostrare politicamente approvando l'ordine del giorno in esame, o diversamente si deve riconoscere che si vuole fare una politica della spesa, come il decreto-legge dimostra. Quindi, o si vuole contenere o si vuole sperperare e purtroppo per acquisire dei voti.

**Il Senato non approva.**

ringrazio il relatore per l'attenzione che ha voluto prestare all'emendamento 1.0.3 chiedendone il ritiro affinché venga esaminato nel disegno di legge relativo al recepimento del recente accordo su lavoro e pensioni. Osservo tuttavia che con ogni probabilità quella legge delega sarà sostituita da emendamenti direttamente prescrittivi che il Governo presenterà al disegno di legge finanziaria, caricandoli con il voto di fiducia, impedendo quindi al Parlamento di esaminare la materia. Si discute molto e giustamente dei bassi salari nel nostro Paese e del loro andamento piatto e moderato nel corso degli ultimi 15 anni. Il tema può essere affrontato concretamente con l'emendamento in esame che è disegnato all'insegna del lavorare di più per guadagnare di più. Quindi insisto nella richiesta del voto. Chiedo che straordinari e premi aziendali vengano così sottratti all'ingiusta progressività che li penalizza; chiedo una sostanziosa detassazione di queste parti

ho sentito dire tantissime volte, da tutte le parti politiche, che bisogna sostenere il reddito ed il potere d'acquisto dei lavoratori. La seconda è che la formulazione di questo emendamento a me pare vada totalmente nel senso di uno dei punti del cosiddetto Protocollo sul *welfare*, in cui le parti sociali ed il Governo hanno concordato di procedere a incentivare, attraverso una minore tassazione, l'orario straordinario, anche perché così emergerebbe una parte del lavoro sommerso. Così ho letto nelle varie stesure, che sono cambiate nei giorni da una parte all'altra; ma questo punto è già lì. Allora, abbiamo oggi l'occasione di cominciare a realizzare un pezzo di quel Protocollo, con l'accordo delle parti sociali, votato da un *referendum* di lavoratori,

dello straordinario e di queste forme di retribuzione, sarebbe francamente un gioco a somma positiva - come si suol dire - per tutti. Per questo motivo, voteremo a favore dell'emendamento

milanese, intasata dal punto di vista del traffico). Sarebbe comunque di per sé una piccola cosa, vista la modesta spesa richiesta, ma un segnale importante per una

tratta veramente di una piccola cosa, che però rappresenterebbe un segnale importante da parte dell'attuale maggioranza verso questo problema settentrionale, di cui tanto si riempie la bocca quando fa i congressi

senatore Baldassarri

Attualmente è in fase concorsuale lo stralcio A del primo lotto, 3° tronco, per 7 chilometri che, verosimilmente, sarà aggiudicato nei primi di gennaio 2008. Il completamento dell'opera è importantissimo, perché essa collega l'Adriatico al Tirreno e per questo occorre una cifra stimata intorno ai 250 milioni di euro. La Regione Lazio ha già stanziato 100 milioni di euro; si chiede al Governo di completare il finanziamento, anche perché ciò risponde a un preciso impegno assunto dal ministro Di Pietro lo scorso anno presso la prefettura di Viterbo.

Le posso garantire che le strade che vanno al di là delle Alpi sono state tracciate da Annibale e da Napoleone. Dunque, abbiamo la necessità profonda di dare respiro ad un'area del Paese, che poi sappiamo mantiene il resto dell'Italia. Vorrei dare un suggerimento gli amici e colleghi della maggioranza, in particolar modo ai senatori del Nord, che ricorderanno sicuramente

queste opere che vergognosamente non sono finite. In particolar modo, chiedo di dare respiro all'aeroporto di Malpensa dove ancora adesso la bretella per il collegamento con l'autostrada Milano-Torino non è stata ancora attuata.

l'emendamento 2.4, sempre per problemi di copertura. Molto spesso non si possono utilizzare gli accantonamenti previsti per i fondi speciali perché sono già stati prosciugati. Quindi, bisogna trovare le coperture all'interno dello stesso decreto

invece, si interviene sui 215 milioni destinati all'ANAS per progetti compresi nel piano di investimenti programmati nel contratto di programma 2007.

Grazie

che ha partecipato nei giorni scorsi ad una riunione promossa dal Presidente della Provincia di Roma, che Enrico Gasbarra ci ha richiamati tutti alla sensibilità perché sul territorio di Roma ci sia una maggiore disponibilità in termini finanziari. il nuovo segretario del Partito Democratico - il sindaco Veltroni - ha promosso analoghe riunioni in Campidoglio, con la presenza di deputati e senatori, sia di maggioranza che di opposizione, richiamandoci alla sensibilità sui temi di Roma, in particolare su quelli che riguardano l'aeroporto di Fiumicino e quindi anche il Comune di Fiumicino, specie alla luce di quanto sta accadendo a livello nazionale, con le relative polemiche che sono nate. Per ultimo ma non ultimo, vorrei ricordare l'accorato appello del presidente della Giunta della Marrazzo che, rivolgendosi ai deputati e ai senatori del Lazio, ha chiesto di intervenire nella sede appropriata, che è questa, al fine di sostenere un impegno diverso per Roma Capitale. In questo senso ci esprimiamo quindi favorevolmente, chiedendo a tutta l'Aula

valga). Su questo provvedimento sono stati presentati qualche centinaia di emendamenti da parte dell'opposizione. Moltissimi di questi emendamenti

localistici e microsettoriali, non basterebbero i soldi, non solo di questo provvedimento, ma dell'intera manovra finanziaria. Comprendo

siamo. Intervengo una sola volta per dire che noi intendiamo mantenere un comportamento rigoroso, ancorché questo dia adito a queste basse speculazioni.

Baccini, e intrattenere brevemente l'Aula sugli argomenti che ha portato nella discussione il senatore Boccia. Il senatore Boccia vorrebbe che l'opposizione rinunciasse a fare il proprio mestiere, cioè proporre argomenti,

perché vedo che da sinistra non c'è nessuna disponibilità, purtroppo non è stato nominato nemmeno un senatore a vita nativo di Fiumicino e, comunque, noi lo approveremo ugualmente. Grazie per la sua disponibilità, Presidente, e per il suo alto tasso di democrazia nel consentirci di parlare.

vorrei però far rilevare al collega Boccia che stiamo discutendo un provvedimento del Governo che ha smaccato carattere elettoralistico, prima di affrontare una finanziaria, che è una finanziaria di spesa, la quale è chiaramente mirata a distribuire denari a Gruppi sociali dei quali si corteggia il favore elettorale. È buona norma all'inizio di una legislatura, quando si pensa di avere davanti a sé un lungo periodo di Governo, imporre agli elettori tutte le medicine amare, ma utili; questo Governo, invece, segue esattamente la procedura opposta: distribuisce denari, evita provvedimenti necessari, ma amari per gli elettori, e dà chiaramente l'impressione di sentirsi prossimo ad una scadenza elettorale e, magari, di tentare di scongiurarla proprio attraverso provvedimenti elettoralistici. Almeno, collega Boccia, ci risparmi una lezione di cui non abbiamo bisogno in materia di integrità.

Presidente, evidentemente si è aperta una ghiotta occasione, che ci è data dal presidente

Come diceva il senatore Storace, basta guardare l'articolo 31, ma non soltanto: è tutto l'impianto di questa legge, che finanzia istituti di ricerca, importanti importanti ricerche scientifiche ed altro, che a volte riescono anche a tenere in piedi in maniera suadente e canuta il Governo, ma ritengo che quanto detto non sia giusto. Per esempio, sono siciliano

compresa la Bindi, hanno avanzato riserve perché non vogliono dotazioni per la Polizia e i Carabinieri, i quali sono colpevoli a Genova di aver massacrato la gente e non di essere stati massacrati, massacrati, colpevoli di non avere la benzina, di avere le macchine vecchie, di non poter perseguire i reati, di non farsi picchiare abbastanza dalla gente, dai *no global* e da altri. Perché non pensano invece, oltre ai fatti particolari, di mettere sulla sicurezza un impegno? Questo impegno ancora ieri è stato disatteso dal Governo Prodi e dal Consiglio dei ministri ed è stato rinviato ancora una volta. Sulla sicurezza la gente è stanca, ma nonostante questo il Governo e parte della maggioranza oppongono un netto no ai rifinanziamenti delle dotazioni dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia di finanza, mettendo in pericolo la sicurezza dei cittadini, che non sono dei particolari, onorevole Boccia, non sono dei microcosmi, ma sono il cosmo perché sono il tessuto di questa Nazione.

Si tratta del cuore della Brianza, che da settant'anni mantiene da sola un altro pezzo d'Italia dieci volte più grande. Se volete dare loro questi 50 milioni per fare un sottopasso ed evitare a chi lavora quattro ore di coda al giorno, fatelo,

agli amici della Lega. Per noi contemporanei, le strade, in Italia, in Europa e quindi nel mondo, le hanno costruite i romani e spesso ci ritroviamo a percorrere le stesse strade dei romani:

Non perseguiamo il medesimo vostro metodo dei noti 1367 commi della vecchia finanziaria per il 2007, da me tecnicamente definiti marchette. Qui si tratta di avere una visione strategica della logistica del movimento di persone e merci nel nostro Paese. Storicamente l'Italia ha una dorsale tirrenica e una dorsale adriatica e altrettanto storicamente non ci sono le trasversali. trasversali. Queste opere, allora, non sono localistiche. Quello illustrato precedentemente dalla collega Allegrini è il completamento dell'asse Adriatico-Tirreno che da Orte porta a Civitavecchia e che collega i due maggiori porti

che non serve per i cisternini o i valmontonesi, ma per dare respiro all'Autostrada del Sole verso la costa tirrenica. Quindi, si può essere favorevoli o contrari, ma non si può definire questa tipologia di emendamenti operette locali territoriali,

che continua a contribuire in modo fuori luogo al bene del Paese stesso, che poi con il cappello in mano deve venire a chiedere

Sentite un po' alle ore 6 di mattina come il Nord del Paese è in coda per poter andare a lavorare, perché non abbiamo strutture, perché viaggiamo - come si diceva prima - sulle strade tracciate da Napoleone e da Giulio Cesare!

come già comunicato durante l'esame del disegno di legge in Commissione bilancio, gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 risultano inammissibili poiché intervengono sui decreti legislativi recanti l'organizzazione e la struttura del Governo. Tali emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 risultano inammissibili poiché intervengono sui decreti legislativi recanti l'organizzazione e la struttura del Governo. Tali emendamenti potrebbero essere, ai fini dell'omogeneità della materia, ripresentati al disegno di legge finanziaria, che, in termini di risparmio di spesa, contiene norme di analoga natura. Passiamo ora all'esame degli

non condivido la decisione assunta dalla Presidenza, sebbene sia consapevole dei limiti regolamentari previsti per i lavori del Senato. avviso, non deve mai confondersi l'assoluta linearità dei comportamenti politici che ci ha indotti, ad esempio, a non considerare l'ennesimo cavallo di Troia che era contenuto nell'ordine del giorno presentato ed illustrato poco fa dal collega Calderoli con l'incapacità di leggere correttamente gli accadimenti, privilegiando la ricerca della verità anche quando comporta un sacrificio. Proprio perché sono convinto che solo gli stupidi

pensando che alcune cose nella vita, anche quando sono sgradevoli, debbano essere accettate ed affrontate. La decisione assunta dalla Commissione bilancio e ribadita poco fa dalla Presidenza con lo *speech* che lei, Vice presidente, ha letto, non risolve il problema del Governo e genera, invece, un doppio danno. I nostri tre emendamenti, signor Presidente (lo dico anche per l'Assemblea), proponevano, con soluzioni diverse, di ridurre la pletorica composizione del Governo. Le soluzioni erano diverse in merito all'efficacia della proposta e valutarle nel merito avrebbe comportato - ritengo - per la maggioranza la possibilità di una disamina corretta. corretta. La soluzione scelta non è condivisibile, perché il decreto-legge oggi al nostro esame è un *omnibus* ordinamentale che si accompagna alla manovra finanziaria, anzi, come diceva ieri il presidente Morando, ne costituisce parte integrante.

sta nella violazione del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, che proibisce l'ingresso in finanziaria

Forse perché qualcuno furbescamente pensa che dopo si potrà risolvere tutto con il voto di fiducia. Ma in questo modo, signor Presidente, potremmo tentare di mettere a posto le carte, dare alla gente quella risposta che che si aspetta e che si aspetta non come vocazione autonoma, ma perché i *leader* di molti grandi partiti della maggioranza, dal neoletto Veltroni al presidente Bertinotti...

al segretario dei Comunisti Italiani, Diliberto, tutti hanno promesso che si procederà in questa direzione. Quindi, raccogliere questa sfida non è una provocazione, ma è un atteggiamento conseguente a valutazioni di carattere politico che sono state fatte dalla maggioranza. dalla maggioranza. Secondo me, con questa scelta la maggioranza e le istituzioni dimostrano, purtroppo, di essere pavide. Ecco perché, signor Presidente, le chiedo un gesto di orgoglio che riscatti almeno le istituzioni, recuperando la correttezza e la trasparenza dei comportamenti, rivalutando la dichiarazione di inammissibilità che è stata formulata testé, proprio perché, applicando il Regolamento, teoricamente questi emendamenti avrebbero diritto di cittadinanza nel decreto-legge, ma non l'avrebbero nella manovra finanziaria. Diversamente Diversamente (ma cercherò fino alla fine, insieme al collega Bordon, di ragionare con la nostra maggioranza e di fare in modo che i comportamenti conseguenti e lineari appartengano a questa grande capacità che ha il centro-sinistra di vivere momenti di diversità e di confusione e poi di recuperare una grande forza per essere consequenziale), mi rassegnerò a discutere in finanziaria questi emendamenti. mi spiace questa rinuncia, che spero però possa vedere una consapevole resipiscenza in un suo comportamento. Qualora non ci fosse, è evidente che inviterò la mia maggioranza ad accettare comunque la sfida, comunque la sfida, che tiene conto di quanto abbiamo detto, sperando che non si debba arrivare a dover chiedere, invece, ad una valutazione numerica dell'Aula l'approvazione di una scelta che tutti facciamo finta di difendere e che dobbiamo avere il coraggio di portare fino in fondo con un atteggiamento che appartiene al DNA che il centro-sinistra ha sempre cercato di mettere in campo. Vi invito a questo senso di responsabilità. Vi richiamo ad una valutazione che sia corretta e consequenziale. Diversamente, la sfiducia di qualcuno di noi non sarà di quest'Aula. Sarà invece una sfiducia che, attraversando il Parlamento, coinvolgerà inesorabilmente i comportamenti di quella gente alla quale quotidianamente ci richiamiamo. Ecco perché, signor Presidente, nell'aspettarmi un gesto dalla Presidenza, voglio che comunque questo momento - che considero infausto - serva alla nostra maggioranza per una presa di coscienza che le faccia comprendere come il mondo fuori di quest'Aula pretenda dei comportamenti concludenti che abbiamo l'obbligo etico, morale e politico di mettere in atto. Mi auguro che ci riusciremo tutti insieme. *(Applausi del

da quello che leggiamo sui giornali; credo però, signor Presidente, che sia diritto dell'Aula sapere in quale fattispecie del Regolamento ci troviamo. Ella ha parlato di inammissibilità. Se non sbaglio, siamo nella fattispecie prevista dagli articoli 126 e 128 del Regolamento, che riguardano l'inammissibilità di emendamenti sui disegni di legge finanziaria e collegati. Se non è questa

nella parte legata alla inammissibilità sulla materia finanziaria c'è una disposizione molto precisa che la Presidenza dovrebbe rispettare. cioè riferimento all'inammissibilità di «emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, [...] che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente»; lo stesso argomento

nell'articolo 97, proibisce di discutere emendamenti che comportano un beneficio per le casse dello Stato. Credo, signor Presidente, che si sia in presenza dell'instaurazione di un precedente pericoloso. che nella comunicazione che ha letto, se l'ho compresa bene, lei ha fatto riferimento alla modifica di un decreto legislativo: ebbene, le ricordo che il decreto-legge, il primo di questo Governo, quello che diede spazio alla spartizione dei Ministeri ed allo spacchettamento degli stessi, era tutto modificativo di decreti legislativi, vorrei capire perché l'Aula non può essere libera di riproporre

possa tornare sui suoi passi e darci la possibilità di discutere; l'Aula poi, con la maggioranza granitica che vediamo, sarà libera di respingere questi emendamenti, ma non si può stabilire un precedente per cui la struttura di governo non si tocca, soprattutto quando ciò farebbe risparmiare gli italiani. punto mi pare di poter dare una risposta definitiva e, come dice ovviamente il nostro Regolamento, inappellabile, perché, non trattandosi di un disegno di legge collegato, valgono le valutazioni che qui ha fatto il Presidente della Commissione bilancio e che sono state sviluppate in quella Commissione. La materia è disciplinata dalla legge finanziaria e del resto lo stesso ordine del giorno G1.100 del senatore Calderoli faceva riferimento precisamente alla legge finanziaria, non al provvedimento oggi all'ordine del giorno.

quindi si aggiunge

Immagino che subito dopo l'Aula voti a favore dell'emendamento 3.0.4, perché proposto dalla Commissione. Tra l'altro, non ho difficoltà a dire che proporrò al Gruppo dell'UDC di votare a favore di quell'emendamento, perché

si rischia di condannare i nostri lavoratori ad avere un trattamento previdenziale più basso rispetto a quello cui potrebbero legittimamente aspirare.

so di certo che, a fronte di un modesto stanziamento di 200 milioni di euro, lo Stato proprio in queste ore risponde invece con un abbassamento delle quote di stanziamento per la sicurezza e per i Corpi di sicurezza (come dicevo prima, Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza). ha un bel dire di guardare alla sicurezza e magari non si agevola la piccola e media industria della Sicilia, che rappresenta uno dei capisaldi importanti per il nostro sviluppo, ma soprattutto per la lotta ai fattori delinquenziali che infestano la nostra terra. in esame. *(Brusìo).* Scusate se interrompo tutti questi conciliabili, però ci sarebbe da prendere atto del parere del relatore sugli emendamenti.

riguarda la modifica delle norme relative alla portabilità del trattamento di fine rapporto, nello specifico interviene eliminando le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Nella norma vi è una dicitura che il senatore Vegas vuole eliminare eliminare perché, per quanto riguarda alcune categorie, alcuni contratti prevedono che ci sia, oltre al TFR maturando che può essere trasferito, anche il contributo aziendale; e giustamente questo contributo aziendale

urlano o parlano contro la delinquenza e a sostegno della piccola e media industria, votare contro l'emendamento che riserva a questo scopo un Fondo, tra l'altro, gestito dal Ministero. Vorremmo vedere le facce dei siciliani quando torneranno a parlare alla Confindustria di Catania, di Palermo, di Messina, di Enna, di Caltanissetta, di Ragusa, di Siracusa o di Trapani. Vorremmo vedere le facce di questi senatori siciliani, quando affermeranno di sostenere la Confindustria e la piccola e media industria siciliana.

Il senatore Strano ha avuto il merito di proporre all'attenzione dell'Aula l'emendamento 3.0.500. Vorremmo sapere se almeno i siciliani che stanno in questo Parlamento siano disponibili ad abbandonare le appartenenze. Su questo emendamento non cade il Governo,

Penso abbia ragione, però purtroppo, come vede, c'è una certa animazione in Aula.

la Campania, ma partecipa al Fondo di solidarietà. Noi la solidarietà la facciamo con 3,43 miliardi di euro,

importante, che ha formato oggetto di attenta analisi della 1a Commissione affari costituzionali. Credo che questa Aula debba licenziare l'articolo 4, se lo riterrà, con le idee chiare anche per chi leggerà poi

prevede la possibilità per il Governo di nominare commissari *ad acta,* previa una procedura di diffida alle Regioni di adottare provvedimenti di natura normativa, organizzativa, amministrativa e così via, entro un termine di 15 giorni.

Quello che però mi preoccupa dal punto di vista costituzionale e istituzionale è che il secondo comma di tale articolo, nel prevedere che in caso di inadempienza il Governo nomini commissari *ad acta*, fa un rinvio al primo comma, dove tra gli atti che le Regioni dovrebbero compiere e che quindi potrebbero compiere i commissari *ad acta* sono previsti anche atti normativi. Tra gli atti normativi vi sono anche le leggi. Credo sia pacifico che i commissari *ad acta* non possano adottare provvedimenti né formalmente né sostanzialmente legislativi. Si va però diffondendo negli ambiti regionali la convinzione e il passaparola che i commissari potrebbero anche sostituirsi ai consigli regionali, ma questa interpretazione è senz'altro esclusa non solo dai lavori della Commissione ma anche dagli interventi svolti in quest'Aula

comma 2, comma superfluo perché stabilisce qualcosa che è già contemplato dalla legge organica sull'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo,

che va proprio nel senso di interpretare la norma in modo univoco, e cioè escludendo che possano essere compiuti atti normativi di carattere generale.

prevede la nomina di commissari per le Regioni inadempienti che sfondano il tetto della spesa sanitaria. L'emendamento 4.1 interviene sulle procedure precommissariamento eliminando la diffida.

4.15, in quanto esso introduce una fattispecie di non eleggibilità per gli assessori, connessa a una scelta di responsabilità oggettiva.

parere conforme a quello del relatore. Colgo l'occasione per precisare che il potere legislativo non è del commissario, mi sembra ovvio.

quel finanziamento scandaloso, rubando dalle tasche degli italiani a cui avete aumentato le tasse per coprire i buchi della sanità portati avanti da Regioni governate da governanti incapaci, avevamo sottolineato alcune questioni. Ad esempio, ogni volta che si

se non li vogliamo mettere in galera e chiedere, come sarebbe giusto, che rispondano almeno percentualmente con il proprio patrimonio dei buchi che hanno fatto con il loro Governo, come minimo siano allontanati per manifesta incapacità di governare.

che le governano, come una volta a chi si macchiava di reati erano tolti i diritti civili, perlomeno per qualche anno si tirino fuori dalla mischia, si riposino, si rinfreschino le idee, vadano a studiare o, magari, cinque anni a lavorare, il che non gli farebbe male, e poi ritornino a fare gli amministratori.

4.9 chiediamo una cosa molto semplice: è ora di finirla che gli amministratori facciano bella figura nella propria Regione con i soldi dei cittadini delle altre Regioni. Non possiamo avere in eterno il Bassolino di turno che spende a destra e a manca, si fa rieleggere con il 70 per cento dei voti perché regala tutto a tutti nella sua Regione, tanto poi i buchi della sua Campania li paghiamo noi della Lombardia.

pagano. I cittadini che per comodità votano il Bassolino di turno, toccati sul portafoglio si renderanno conto di quello che i propri amministratori fanno e la volta dopo non li voteranno più, se non volete toglierli già d'ufficio dal loro posto; posto; se oltre un certo limite devono tirare fuori i soldi dalle loro tasche, forse entreranno nell'ordine di idee che è meglio chiudere la sede a New York della Regione Campania,

a coprire con i soldi degli altri i propri buchi, spendono soldi non propri, ma ne spendono di più. Non è che la Regione Campania faccia un buco perché i campani non pagano le tasse, però però almeno spendono meno soldi, no: le Regioni Campania, Calabria e Sicilia spendono 150‑200 euro in più all'anno per abitante e in aggiunta ne fanno altrettanti di buco, tant'è che alla fine siamo qui sempre ogni volta a coprire questi buchi. Quindi, veramente,

perché se è giusto introdurre dei meccanismi di responsabilizzazione delle Regioni che sforano i parametri della spesa sanitaria, è assolutamente ingiusto aumentare ancora la pressione fiscale,

Invece, le Regioni devono essere responsabilizzate principalmente sul comparto della spesa. Devono quindi essere precisati e migliorati i meccanismi di contenimento della spesa, piuttosto che scaricare su una fiscalità che in questo Paese è già fin troppo eccessiva per demerito, penso, dell'attuale gestione del sistema fiscale.

Dichiaro aperta la votazione.

È chiaro che siamo assolutamente contrari all'incremento della pressione fiscale ma qui, visto che siamo a Roma, è ora di finirla di parlare del pollo di Trilussa.

la sanità che non fa i buchi e coprono i buchi degli altri. Se alla Campania aumentiamo di 50 euro per famiglia o per persona l'IRAP, così mandano a casa Bassolino, credo sia un investimento per tutta la Nazione, non un incremento della pressione fiscale. Se l'IRAP, che dovrebbe andare a coprire gran parte della sanità, viene pagata per l'85 per cento sopra al Po, questo, senatore Vegas, è un problema da risolvere non solo per la Padania ma per l'Italia,

per il compimento degli atti di cui al primo comma dello stesso articolo 4 nel quale sono indicati anche "atti normativi", ritenuto che da una lettura superficiale potrebbe desumersi che i commissari governativi possano approvare anche atti legislativi; considerato peraltro che il sistema delle fonti riserva in via tassativa con inequivoche norme di rango costituzionale la potestà legislativa solo ai Consigli regionali ed al Parlamento nazionale secondo le rispettive competenze,

perché l'arbitraria definizione di rarità non ha agevolato assolutamente la ricerca. Pertanto, aiutare le ditte farmaceutiche che producono questi farmaci orfani, per malattie che

di quelli preventivati, il *budget* regionale splafona e normalmente queste persone incontrano grandissime difficoltà nel reperire questi farmaci che, tra l'altro, sono costosissimi. Ci sono Regioni

Se istituissimo un centro di riferimento, un centro di costo nazionale, potremmo bypassare la problematica regionale e dare copertura finanziaria a questi pazienti, perché oltre alla malattia rara

perché, non avendo un registro nazionale, non sappiamo esattamente quante sono le malate, dove sono allocate e dove, di conseguenza, indirizzare le risorse nei centri di riferimento.

l'altro, presso l'Istituto superiore della sanità è già previsto un registro sulle patologie di infertilità e il 30-35 per cento di malate di endometriosi - stiamo parlando di una donna su dieci

Attualmente l'attribuzione del ripiano dell'eventuale sfondamento della spesa farmaceutica territoriale è affidata per il 100 per cento a carico esclusivo della sola filiera. della sola filiera. Questa attribuzione risulta a nostro avviso inaccettabile perché, da un lato, le imprese farmaceutiche hanno l'obbligo di fornire, ma, dall'altro,

proposto in materia di regolazione dei prezzi dei farmaci, e al mantenimento del prezzo di riferimento sui soli prodotti a brevetto scaduto, così come è già stato definito dall'AIFA. Nella motivazione del documento del tavolo si indicava il rischio di una disomogeneità del sistema di regolazione dei prezzi da Regione a Regione e della perdita di una sorta di coerenza del sistema di regolazione nazionale. Conla modifica del regime di controllo della spesa farmaceutica territoriale verrebbe a cadere ogni ragione perché debba continuare a sussistere una norma come quella dell'articolo 10 della legge n. 405 del 2001, sul prezzo di rimborso di particolari categorie di farmaci in relazione potrebbe essere davvero distorsiva del mercato e disincentivante dell'attività di ricerca. Per questo riteniamo opportuno abrogare esplicitamente la norma suddetta. La ragione dell'emendamento 5.45 5.45 nasce dal tentativo di impedire aumenti eccessivi in una volta sola. Infatti, per effetto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 149 del 2005, il prezzo dei medicinali non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale

Questa disposizione comporterebbe il rischio di aumenti consistenti concentrati in un unico mese, ogni due anni. Perquesto riteniamo che sarebbe necessario rivedere la norma consentendo la modifica in aumento ogni anno, magari entro il mese di gennaio, stabilendo un tetto massimo pari al tasso di inflazione, salvo ovviamente casi eccezionali che dovranno essere opportunamente motivati dalle aziende all'AIFA. Una norma di questo genere consentirebbe di evitare brusche variazioni dei prezzi dei farmaci non rimborsabili ogni due anni, con effetti negativi anche presso l'opinione pubblica.

un parere su questi emendamenti, tuttavia l'orientamento del relatore e del Governo è di concentrare l'attenzione, rispetto a tutta questa partita, su un problema che avevo già anticipato nella mia relazione, quello cioè di intervenire trovando le risorse adeguate - lo stiamo ancora facendo, non lo dico per rinviare il problema, ma perché ci stiamo lavorando

alla senatrice Bianconi di ritirare i suoi emendamenti, che affrontano problemi di grandissima importanza, ma per i quali non siamo in grado in questo momento di trovare le coperture adeguate.

è stato uno dei fondatori della Regione Marche dove ha ricoperto gli incarichi di Capogruppo della Democrazia Cristiana e più volte assessore. È stato anche Sottosegretario alla sanità nel II Governo Craxi e nel VI Governo Fanfani e Sottosegretario ai lavori pubblici nel Governo Goria. *Leader* della DC picena e marchigiana, è stato protagonista degli anni della ricostruzione. Espressione della realtà popolare, ha rappresentato gli interessi sociali e culturali del popolarismo cattolico. Sono cresciuto politicamente con lui nella DC e di lui ricordo il rispetto politico e umano degli avversari politici che hanno rappresentato, per diverse generazioni politiche della Democrazia Cristiana, una scuola politica e umana improntata ai valori della democrazia e del cristianesimo. Esprimo, anche a nome dell'UDC, le più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie Italia, ai figli Alessandra, Giorgio,

si associa alle parole pronunciate dai senatori Ciccanti e Baldassarri per il lutto che ha colpito la famiglia Nepi nella persona del senatore Gualtiero Nepi.